La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha adottato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 7 giugno 2007. Resta confermata per oggi pomeriggio la discussione del disegno di legge concernente i cognomi dei coniugi e dei figli. Sarà inoltre inserita all'ordine del giorno odierno la ratifica dell'Accordo internazionale con Israele in materia di navigazione satellitare. Il calendario della settimana è poi integrato, a partire da domani, con il disegno di legge recante interventi contro lo sfruttamento di lavoratori stranieri clandestini, per il quale il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 di oggi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi. Resta poi confermato per la settimana corrente l'esame della delega in materia di liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas. Sempre nel corso di questa settimana, il Parlamento in seduta comune è convocato, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, domani alle ore 14 e giovedì 31 maggio alle ore 10. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. Rimane confermata, giovedì pomeriggio, la seduta per il sindacato ispettivo. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, la seduta pomeridiana di martedì 5 giugno si aprirà con la deliberazione, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, sull'urgenza dell'affare inerente la revisione delle leggi elettorali, avanzata dal senatore Calderoli. Il calendario della prossima settimana prevede poi l'esame delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro e di riordino dei servizi pubblici locali. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 6 giugno, sarà discussa la mozione Schifani ed altri sulla revoca delle deleghe al vice ministro Visco congiuntamente ad altri connessi strumenti, anche di sindacato ispettivo.

per le medesime motivazioni per cui, in chiusura dei lavori prima della sospensione per le elezioni, avevamo proposto come elemento fondamentale di discussione la delega sulla liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas, e quindi tutte le questioni inerenti a questi rilevanti

trasmissione dei dati della relazione trimestrale dell'ARAN. Come lei sa, si tratta di dati che il Parlamento deve costituzionalmente avere. Oggi abbiamo appreso dalle agenzie che è stato concluso un ulteriore accordo tra i sindacati e il Ministro per le riforme e le è il terzo accordo che si raggiunge senza che il Parlamento abbia dei dati essenziali per poter espletare la sua funzione di controllo. Abbiamo sollecitato il Governo in questo senso con un'interrogazione.

solo due brevi considerazioni aggiuntive. La prima è che la Commissione giustizia ha iniziato l'esame dei disegni di legge in materia, d'iniziativa parlamentare, il 19 settembre, vi ha dedicato otto sedute e ha approvato il testo il 17 gennaio, a maggioranza. La seconda considerazione è la seguente: la necessità di legiferare in materia discende da una sentenza della Corte costituzionale - tutto ciò è nella relazione scritta, per chi vorrà leggerla - che ha ritenuto essere costituzionalmente illegittima, per la disparità di trattamento esistente tra uomo e donna, tra marito e moglie, l'attuale disciplina del cognome famigliare e ha ritenuto tuttavia, per la pluralità di scelte di metodo che possono essere adottate al riguardo, di tradurre quest'affermazione in una sollecitazione al Parlamento ad intervenire.

come le stesse legislazioni europee - che hanno quasi tutte (dalla Francia, alla Germania, alla Spagna) legiferato in questi anni in tal senso - dimostrano, avendo adottato soluzioni paritarie quanto agli effetti, ma non identiche quanto alla struttura. Pertanto, il relatore e la Commissione sono disponibili, qualora si dovessero trovare soluzioni più persuasive e dotate di più ampio consenso parlamentare, a ritenerle valide. In particolare, tra gli emendamenti che sono stati presentati, a me pare (e forse non solo a me) di un certo interesse quello che vede come primo firmatario il senatore Valditara. Tuttavia, al di là di queste considerazioni, il dato che mi premeva sottolineare

non ci sono soluzioni rigidamente precostituite, ben consapevoli che quella prevalsa in Commissione è una delle possibili soluzioni da adottare. Per il resto, mi rimetto alla relazione scritta.

non solo in ragione della nostra Costituzione ma anche per profonda convinzione, noi riteniamo che il Parlamento sia il luogo dove non solo si parli per esprimere un'opinione, ma si ricerchi tra maggioranza ed opposizione ogni possibile convergenza. Nel nostro programma abbiamo sottolineato che sulle grandi questioni istituzionali, sulle riforme di sistema e su quelle che riguardano l'organizzazione e la vita della comunità non avremmo proceduto con votazioni a maggioranza.

Anzi, vorrei annunciare che parteciperemo alla discussione dopo aver chiesto ai colleghi di esprimere liberamente le proprie posizioni. Abbiamo già chiesto al presidente Salvi, che è anche relatore del provvedimento, di farsi carico delle nostre posizioni e di quelle dei colleghi del centro‑destra, affinché su questa materia si realizzi una grande convergenza. Signor Presidente, è un tema importante e per qualche verso

di esprimere in un dibattito parlamentare che non può che risultare costruttivo. Pertanto, signor Presidente, condivido pienamente l'impostazione data dalla Conferenza dei Capigruppo e che lei ha richiamato;

perché lei rubrica la questione avanzata dal collega Franco Paolo come una proposta della Lega? Io la ritengo una proposta di grande buon senso e cercherò di spiegarlo, posto che probabilmente in tutti i Gruppi ci sono dubbi e perplessità a favore o contro; quindi, sarà un tema che probabilmente vedrà una trasversalità nell'espressione del voto. Tuttavia, presidente Marini,

Ecco perché vorrei un soprassalto di ragionevolezza. Visto che si dice che questo testo probabilmente dovrà essere rimaneggiato, non sarebbe meglio discuterne in Commissione per portare qui il testo su cui si vuole affrontare

dignità, che il Senato ha già preparato e discusso lungamente in Commissione e che è da parecchio tempo all'attenzione anche della Conferenza dei Capigruppo

Nel momento in cui, però, lei entra nel merito, in qualche modo, influenza il giudizio e ne fa una valutazione «di parte». Noi abbiamo posto semplicemente una questione sospensiva

Il Senato non è in numero legale.

Signor Presidente, ritengo opportuno e giusto discutere di questo argomento. Capisco le esigenze esistenti, capisco ci siano anche aspettative, ma certo - sono d'accordo con chi l'ha detto prima - non la reputiamo una priorità. Oltretutto, se vediamo nello specifico questo disegno di legge, possiamo solamente giudicarlo dispersivo, se vogliamo essere gentili, perché andrebbe definito confusionario; dispersivo perché strutturato in questo modo porta solamente alla dispersione... è dispersivo perché, strutturato in questo modo, porta solamente alla dispersione della nostra storia, della nostra tradizione e della nostra cultura che volenti o nolenti, sul grande e indispensabile nucleo della famiglia. Con questo provvedimento non si capisce cosa possa succedere: tutto è permesso, non ci sono idee, non c'è una guida politica.

che trovano la maggioranza totalmente divisa e in stato confusionale. Aspettiamo, signori del Governo, la discussione sui DICO. Mi pare che la Conferenza convocata dal ministro Bindi non abbia fatto altro che aprire crepe; credo proprio che quello che teme la maggioranza sia che di crepe se ne aprano tante altre perché, come abbiamo visto, da essa non è scaturito proprio nulla di nuovo. La grande manifestazione del *Family Day* ha preoccupato molti della maggioranza, che ora non sanno più cosa fare. Anche per questo riteniamo sia assolutamente sbagliato procedere su una strada lastricata solo di demagogia e di propaganda. Noi siamo pronti, invece, a lavorare per trovare un'intesa e accogliamo con favore la disponibilità oggi dimostrata dal presidente Salvi. Rinviamo dunque il provvedimento in Commissione e, senza sconvolgere l'istituzione famiglia, diamo finalmente un segnale che questa politica ha voglia di rispondere ai veri problemi delle famiglie italiane e che su questi problemi siamo capaci di unire.

e ai proponenti della scorsa legislatura, come a quelli della presente, esso sembrerebbe trovare giustificazione e traccia, oltre che nell'articolo 3 della nostra Costituzione, in precedenti deliberazioni sia della Corte europea che in un Trattato stipulato a New York nel 1978 e ratificato nella legislatura precedente.

dato a scelta, senza che esso sia quello del padre o della madre. Diciamo, quindi, che in Europa si è generato un sistema giuridico quasi da *discount* del cognome e che questo sia un fatto non solo di scelta, ma di opinabilità. Io personalmente e noi come Gruppo siamo assolutamente contrari a quanto, di fatto, è stato superato dalla storia e dalla tradizione. Infatti, la nascita dei cognomi si ha nel secondo medioevo quando, con il riconoscimento e la registrazione avvenuta dopo il battesimo negli archivi ecclesiastici, si poneva,

il calzolaio negli altri linguaggi europei, superava una difficoltà della tradizione del diritto romano secondo cui bisognava ricorrere, per identificare il nuovo nato, non soltanto al nome del padre e della madre, ma anche a quello della *gens*. Questo sistema immediato, concreto, naturale, viene dato nei tempi bui, nel secondo medioevo, attraverso l'abbinamento del cognome e con l'identificazione del nuovo nato, per esempio, con un artigianato e cioè con un modo di essere, un modo di fare, con una tradizione propria, e quindi, contrariamente a quella che poteva essere ipotizzata una ribellione dei popoli sottomessi, i franchi, i bretoni e gli ispanici, mentre questi oggi si rifanno ad una tradizione che avrebbe dovuto, per loro antica sottomissione, essere contraria al diritto romano, vogliono complicare il modo molto più semplice e agevolato nato nel secondo medioevo, riconducendosi ad una varietà di possibilità di attribuzione del cognome che è quella superata nel secondo medioevo, tradizione nella quale noi invece ci riconosciamo perché è quella più immediata

dall'ordine alfabetico. A questo punto vedremo che chi non si riconosce in questa necessità cercherà di sposarsi, se si chiama Agnello, con chi si chiama Zullo, Zucchero o Zuzzurro, e dunque chi nel giudizio universale

dell'altro coniuge, che magari si chiama Adamo, Agnello o Amore. Al di là di queste osservazioni specifiche, ve n'é un'altra un'altra che avrebbe potuto essere trattata probabilmente con una pregiudiziale che ci trova assolutamente contrari, ed è la difficoltà che questo disegno di legge, se approvato, introduce nel nostro ordinamento e specificamente nell'ordinamento degli enti locali. Dico questo nella precedente legislatura, una delle osservazioni che fu fatta in Commissione bilancio e che non fu possibile superare era quella del costo dell'introduzione di una sistematica di questo tipo. Infatti, se se ci sono due genitori che scelgono di dare al figlio, all'interno del matrimonio, un cognome - visto che lei, mi permetta Presidente, è uno dei pochi che mi sta a sentire

il secondo figlio non può chiamarsi Malan Ferrara, ma dovrebbe chiamarsi Ferrara Malan. Affinché ciò possa essere accertato e ricondotto alla sistematica, come disposto dal disegno di legge, bisognerebbe far sì che la

questione del doppio registro è semplice da raccontare. I registri dei nati vengono conservati in due luoghi diversi sin da quando, durante i primi moti dei fasci di combattimento, i municipi vennero assaltati

gli enti locali e l'Associazione dei Comuni hanno affermato che ciò non è assolutamente vero. È allora molto più plausibile credere che sia ancora valida la riserva del Ministero dell'interno

così tanti lustri per poterne parlare perché l'articolo 3 ha certamente tanti significati, ma non specificatamente quello che si vuol considerare come presupposto e ipotesi per costruire la tesi del disegno di legge Al di là di queste dissertazioni, per quello che mi compete e per quello che ho vissuto in Commissione bilancio nella precedente legislatura e in questa, il provvedimento è sicuramente contrario alla Costituzione perché non contiene alcuna previsione di costo e quindi nessuna copertura relativa,

che chiaramente si è approcciato in modo molto economico - se mi si passa il termine - alla tematica, che non ha soltanto i riflessi Preliminarmente, nell'affrontare la normativa sottoposta alla votazione dell'Assemblea, occorre considerare che essa tende innanzitutto a realizzare quel principio di eguaglianza fra uomo e donna, rispetto al vincolo matrimoniale e alla filiazione, in attuazione sia dei princìpi costituzionali, sia di numerose pronunce in sedi internazionali, sia infine recependo... - se il relatore mi dà un'opportunità, dato che siamo così pochi in Aula

alle indicazioni della Corte costituzionale - giusto perché resti agli atti con puntualità il riferimento - chiaramente intendo operare un confronto con la sentenza del 6 febbraio 2006, n. 61, con la quale il giudice delle leggi ha sottolineato come l'attuale sistema di attribuzione del cognome sia un retaggio di una vecchia concezione patriarcale della famiglia e di una ormai tramontata potestà maritale, entrambe non più coerenti con i princìpi dell'ordinamento, con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna e con i vincoli e gli stimoli provenienti dalle fonti del diritto internazionale. La normativa al nostro esame, per semplificare il problema, affronta due diversi profili: da una parte, quello relativo al cognome della donna coniugata; dall'altra, quello relativo al cognome dei figli. Per quanto riguarda il primo,

l'articolo 143-*bis* del codice civile, nel senso che ciascun coniuge possa conservare il proprio cognome. Tale abrogazione riflette la precisa volontà di completa rimozione dal nostro ordinamento di ogni traccia dell'istituto della potestà maritale. L'aggiunta del cognome del marito a quello della moglie, secondo quanto previsto dall'articolo 143-*bis*, si giustificava - non voglio usare il presente perché ritengo che, di fatto, questa sia una norma non più utilizzata - nella prospettiva di preminenza del marito rispetta alla moglie. Considerando, però, l'esperienza attuale italiana, va osservato come nell'esercizio della loro professione e di tante altre attività molte donne oggi, di fatto, evitano di servirsi del doppio cognome presentandosi unicamente con la propria identità. Nella sostanza, in quasi tutte le situazioni giuridicamente rilevanti dal punto di vista amministrativo, civile o fiscale, il cognome che viene in considerazione per le donne coniugate è quello di nascita, anche in conseguenza dell'ormai prevalente utilizzazione in tutte le sedi del codice fiscale, come ci ricordava il Governo in Commissione, che come noto non viene modificato in seguito al matrimonio. Quindi, quella previsione del codice viene puntualmente smentita laddove, per esempio, il codice fiscale non risente assolutamente di quella norma. L'aggiunta del cognome del marito ancora oggi, piuttosto che essere un simbolo dell'unità della famiglia, resta simbolo di tali ancestrali concezioni, rappresentando ancora un segno di appartenenza incompatibile con il precetto costituzionale di parità dei coniugi. Quindi, la prima parte della puntuale proposta normativa sottoposta all'esame dell'Aula è assolutamente condivisibile, laddove prevede l'abrogazione dell'articolo 143-*bis*. Per la verità, e questo appunto viene ripreso da un mio emendamento, il disegno di legge all'esame dell'Aula prevede la modifica dell'articolo 143-*bis*, nel senso di

prevedere che la donna fosse "obbligata" ad aggiungere il cognome del marito nel momento in cui si sposava. Comunque, rispetto a questa parte dei disegni di legge - infatti in tutte e tre le proposte presentate in Commissione giustizia si prevedeva la stessa cosa si può tranquillamente dire che c'è una sostanziale condivisione, al di là del fatto se si modifica l'articolo 143-*bis* o, invece, come faccio io, se ne propone l'abrogazione poiché, obiettivamente, è una norma che non serve più.

alla seconda questione affrontata dal provvedimento, quella del cognome dei figli. In questo caso caso dobbiamo considerare che la proposta della Commissione è quella di lasciare ai genitori la possibilità di attribuire o il cognome del padre o quello della madre o quello di entrambi, salvo disaccordo, nel qual caso l'ufficiale di stato civile attribuisce al nato i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, tutto ciò facendo salvo il mantenimento dei cognomi attualmente attribuiti. La proposta contenuta nell'articolo 2 è stata oggetto di un mio emendamento, sulla base di considerazioni che ci sembrano abbastanza semplici: perché attribuire la facoltà di dare solo il cognome del padre o solo il cognome della madre, aumentando la confusione, la possibilità di liti e di disagio sociale conseguenti alla novità? Perché costringere la gente a dibattere e a scegliere quando è possibile un tranquillo automatismo, quello indicato nel mio emendamento? Se il senso è quello di ragionare su un rapporto che tocca il minore, che non appartiene più al padre né alla madre,

significato nel momento in cui automaticamente prevediamo che entrambi i cognomi entrino nel patrimonio genetico e sostanziale del neonato. Altrimenti, daremo la stura a una serie di problemi che innanzi all'ufficiale dello stato civile

si rafforza quella bigenitorialità, si rafforza quella circostanza che di fatto invece mancherebbe e cioè che il figlio è di entrambi. In tal modo, proprio nell'interesse del minore, si verrebbero a

entrambi, che produrrebbe un meccanismo farraginoso, che personalmente mi sembra più foriero di ulteriori problemi che non di una soluzione di quelli all'ordine del all'ordine del giorno. É quasi come se - e mi avvio a chiudere, Presidente - ci fosse una proposta monca, laddove, da una parte, condividiamo la necessità di liberarci di vecchi orpelli che appesantiscono appesantiscono la nostra legislazione, dall'altra, non abbiamo però il coraggio di compiere fino in fondo una scelta che invece merita, se condivisa, di essere portata tranquillamente avanti. Ecco perché il mio mio parere sarebbe quello, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, di ragionare sulla possibilità di rivisitare la normativa che abbiamo proposto all'Aula,

l'ipotesi di un ritorno in Commissione non venisse condivisa da tutti gli oratori e da tutti i Gruppi, continuerei a sostenere gli emendamenti che ho proposto, che sono emendamenti per qualche verso completamente sostitutivi, che però non avrebbero l'avallo di una discussione precisa e puntuale, che invece in Commissione può essere ancora recuperata.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, penso che un ringraziamento alla Commissione giustizia per essersi fatta carico di un'iniziativa legislativa parlamentare per la nuova disciplina del codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli sia giusto e doveroso. Come ben si comprende, due sono i profili giuridici presi in considerazione; il primo è il cognome dei coniugi, il secondo è la trasmissione ai figli del cognome dei genitori. Com'è stato osservato, allo stato delle cose, nel nostro ordinamento, non esiste una norma che disciplini espressamente l'attribuzione del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio, ma tale osservazione vale anche per i figli naturali nati fuori dal matrimonio. Sta di fatto che, per inerzia, si è conservata la prassi della potestà maritale dell'*ex* articolo 144 del codice civile precedente la riforma del diritto di famiglia del 1975. Come rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 12 febbraio 2006, l'attuale sistema maritale non è coerente con l'articolo 3 della Costituzione, che prefigura appunto un'eguaglianza sostanziale tra i sessi. Parimenti, la Cassazione, con ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004,

Infatti, per ragioni amministrative, previdenziali, sanitarie e giudiziali, il problema del cognome maritale per il coniuge si pone senza eccessivo impatto, perché il cognome identificativo della donna è sempre quello anagrafico, quindi il problema in qualche modo si risolve da solo sotto quest'aspetto; basti pensare che il codice fiscale riassume i dati anagrafici originari della donna e che tale identificazione fiscale rappresenta oggi anche un'identificazione informatizzata, giuridicamente rilevante in tutte le piattaforme digitali che caratterizzano la pubblica amministrazione. Quello che riverbera in modo significativo dell'esigenza di eguaglianza tra uomo e donna è l'attribuzione del rispettivo cognome ai figli. Tale problematica è stata affrontata, negli ultimi anni, da numerose legislazioni europee, alcuni esempi. In Spagna, il figlio assumeva il doppio cognome, quello paterno seguito da quello materno, con trasmissione di quello paterno alle generazioni successive; nel 1999 si è stabilito, invece, che tale automatismo dovesse cedere il passo all'accordo tra i coniugi su quale cognome, appunto, trasmettere alle future generazioni; in mancanza di accordo, prevale il cognome paterno, denunciando, pertanto, una sostanziale ineguaglianza tra i sessi. In Germania, si può scegliere con quale cognome identificare la famiglia; in mancanza di accordo, ciascuno può conservare il proprio cognome, in quest'ultima ipotesi, si concorda, all'atto della nascita del primo figlio, quale dei due cognomi trasmettere al figlio. In Francia i genitori si accordano su quale cognome dare ai figli, ovvero si attribuiscono entrambi i cognomi nell'ordine concordato:

In Gran Bretagna prevale la stessa disciplina della Francia: in Galles e in Inghilterra, però, si può addirittura scegliere un altro cognome, diverso da quello dei genitori. In Italia si sarebbe potuto procedere in più direzioni prevedendo, innanzitutto, il doppio cognome obbligatorio con opzione legale o volontaria sull'ordine dei cognomi, per i figli nati nel matrimonio;

ovvero del figlio, se ha compiuto 14 anni. Sul primo aspetto, l'articolo 143-*bis* del codice civile viene modificato nel senso che al figlio è attribuito il cognome del padre o della madre, secondo accordo, ovvero tutti e due i cognomi dei genitori. Con quale ordine? L'ordine è importante perché poi il figlio trasmetterà al proprio figlio il primo cognome.

Se c'è accordo, il problema si risolve da solo. Se l'accordo invece manca, per garantire il principio di uguaglianza, nel senso che l'uno e l'altro cognome hanno pari priorità, si è decisa l'opzione legale, a dire che la registrazione anagrafica è in ordine alfabetico. Qualcuno aveva proposto il sorteggio, qualcun altro il primo cognome, quello della madre, quale cognome naturale che precede addirittura la nascita. Da uomo e da padre egoisticamente avrei preferito una soluzione come quella spagnola o francese, cioè mantenere il primo cognome paterno in caso di disaccordo. È prevalsa, invece, la tesi di un'uguaglianza sostanziale tra i coniugi, in caso di mancato accordo, e onestamente la condivido. Sta di fatto, però, che i genitori decidono in via prioritaria come comportarsi all'atto del matrimonio, cioè nella fase più serena del rapporto e delle valutazioni sociali, economiche, religiose e sentimentali: quindi sceglieranno sicuramente nell'interesse del figlio. A maggior ragione, se la scelta è rimessa al momento della nascita, perché in tale occasione la centralità del figlio è prevalente su quella degli interessi o dell'orgoglio di uno dei genitori. Rimane il problema irrisolto della trasmissione del cognome ai figli nati dopo il primo, se questo è nato prima del matrimonio. La casistica che si riscontra in queste circostanze è ampia e a volte, troppe volte, con forti condizionamenti psicologici in merito al problema del riconoscimento di paternità. In tal caso, se non c'è un accordo, il potere di interdizione dell'uno o dell'altro dei genitori può essere più decisivo degli interessi dei figli futuri. Rimane, inoltre, anche il problema del vincolo per il figlio di un cognome indesiderato, che può essere tale per molte ragioni (giudiziarie, morali, economiche, personali): doverlo accettare come un marchio è un limite non rimosso dall'attuale disegno di legge. Non sarebbe stata scandalosa la facoltà di cambiare cognome, come avviene in Inghilterra. Anche adesso in Italia si può cambiare cognome, ma con una procedura burocratica lunga e farraginosa, dove la libertà dell'individuo è rimessa alla discrezione del burocrate, dell'autorità amministrativa, quando questa facoltà dovrebbe essere lasciata, indipendentemente dalle valutazioni burocratiche, alla libertà del singolo. La famiglia è una cosa diversa dal familismo. Sta il fatto, comunque, che l'articolo 2, comma 5, del disegno di legge così come proposto dal relatore in Commissione - stabilisce che il figlio a cui sono stati attribuiti dai genitori entrambi i cognomi è poi libero di scegliere quale dei due trasmettere al proprio figlio. Questa norma risolve molte questioni - non tutte - rispetto a quelle dianzi sollevate. Positiva è inoltre la scelta dell'articolo 6 di anteporre al cognome dell'adottato quello dell'adottante che segue la dinamica del cognome dato ai figli nati nel matrimonio. Infatti, mi sembra giusto che all'adottato non sia tolto, se l'ha, il proprio cognome, senza con ciò ignorare quello dell'adottante che gli ha dato una nuova famiglia. Risolvere il problema imponendo il solo cognome di uno di tutti e due i nuovi genitori potrebbe significare la cancellazione di un'identità condivisa, imponendo la volontà di una parte su quella più debole. Su questo disegno di legge di modifica della disciplina dei cognomi nel codice civile si è aperto un confronto a più ampio raggio, vedendoci qualcuno anche un indebolimento dell'istituzione famigliare. Sicuramente una visione tradizionale della famiglia - per intenderci, quella fondata sul *pater* *familias* - è però decisamente superata. Ciò non significa che la famiglia moderna, fondata sulla responsabilità di ambedue i coniugi, quella costituzionale dell'uguaglianza dei sessi, quella del nuovo diritto di famiglia, fondata più sulla genitorialità che sulla coppia, che implica una donna che lavora e assume, pertanto, gli stessi obblighi e doveri del marito in ordine al mantenimento e all'educazione dei figli,

Certo, la famiglia ha bisogno di ben altre e più importanti riforme. Aspettiamo con ansia politica per discuterne e in tal senso sollecitiamo il Governo e la maggioranza. Un'ultima considerazione: credo che debba essere accolto l'emendamento 8.3, a firma del presidente D'Onofrio, che propone il 1° gennaio 2008 quale data di entrata in vigore della legge, per lasciare un congruo lasso di tempo per prepararsi (anche culturalmente) a tale rilevante cambiamento di costume della famiglia italiana. Per tutte queste ragioni, condivido nel complesso il disegno di legge in discussione, salvi i miglioramenti possibili per i punti di criticità

Signor Presidente, signori senatori, sono passate appena due settimane dalla manifestazione che si è svolta a piazza San Giovanni: una straordinaria mobilitazione popolare che ha inteso riaffermare il ruolo fondamentale e centrale della famiglia all'interno della società italiana. In quella occasione più di un milione di cittadini è sceso in piazza per reagire contro gli attacchi che alla famiglia vengono rivolti in maniera sempre più frequente, ma soprattutto per sollecitare una sua tutela a livello giuridico oltre che a livello economico. Piazza San Giovanni è stata il grido della società cattolica e della società laica a favore della famiglia. Ebbene, anche traendo spunto e vigore dalla volontà manifestata in maniera inequivoca dal popolo italiano lo scorso sabato 12 maggio, oggi esprimo le mie perplessità rispetto al disegno di legge che siamo chiamati a votare. Esso, lungi dal voler affrontare le situazioni di reale disparità che ancora sono presenti nel codice civile, si risolve nei fatti nell'ennesimo subdolo attacco alla certezza che l'istituto della famiglia porta con sé. Leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, vediamo richiamata, quale giustificazione delle novelle introdotte, una sentenza piuttosto recente della Corte costituzionale, la n. 61 del febbraio 2006. In essa, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulle disposizioni codicistiche in materia di cognome dei coniugi e dei figli, riconosceva la necessità di una rivisitazione della materia, muovendo dalla considerazione che l'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e col valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. La Corte costituzionale rimetteva perciò al legislatore e alle sue valutazioni politiche il compito di procedere alle necessarie operazioni Ebbene, leggendo il disegno di legge in esame, ci rendiamo conto che tra tutte le opzioni percorribili per ottemperare alla pronuncia della Corte è stata scelta quella peggiore, che ha sostituito ad un sistema di individuazione certo e sicuro un sistema del tutto casuale ed anarchico, che genera enorme confusione e dunque una grossa conflittualità. In particolare, l'articolo 143-*bis*.1, che introduce *ex novo* nel codice la disciplina del cognome del figlio di genitori coniugati, fino ad oggi frutto di consuetudine, appare estremamente confuso e censurabile. Manca, infatti, un criterio chiaro ed univoco di individuazione di tale cognome, ben potendo essere il solo cognome della madre, il solo cognome del padre oppure quello di entrambi nell'ordine da essi stabilito o in ordine alfabetico in caso di disaccordo. Nulla si dice, peraltro, delle ipotesi in cui padre e madre abbiano già due o più cognomi ciascuno, cosa che potrebbe avvenire assai frequentemente in futuro, nella malaugurata ipotesi che questo disegno di legge fosse trasformato così come è in legge. Insomma, se lo scopo del diritto è quello di disciplinare rapporti giuridici meritevoli di tutela, in modo da assicurare certezza ad essi, prevedendo e risolvendo possibili ragioni di conflitto, il risultato che questo disegno di legge consegue è esattamente l'opposto. Si sostituisce ad un sistema certo un sistema incerto, casuale e dunque potenzialmente conflittuale: non ne vediamo davvero la ragione. Raccogliere il monito della Corte costituzionale avrebbe richiesto ben maggior coraggio di quello dimostrato dagli autori di questo disegno di legge, che si sono limitati a rimettere al libero arbitrio dei coniugi la scelta di un elemento fondamentale quale il cognome di un figlio, che individua l'appartenenza dell'individuo ad una famiglia, cioè alla più importante comunità sociale, fonte di obblighi e diritti insostituibili. Se il disegno di legge verrà approvato senza modifiche, tra qualche anno non solo i figli di fratelli, ma anche nonno e nipote o padre e figlio potranno avere cognomi diversi e l'effetto perverso sarà quello di perdere l'elemento di identificazione che contraddistingue gli appartenenti alla stessa famiglia, e questo non è solo un fatto burocratico e formale, in quanto la famiglia è portatrice di un irrinunciabile patrimonio culturale, di tradizioni, in definitiva del nostro vissuto. Bene e meglio si poteva fare per coniugare i princìpi di uguaglianza tra i coniugi e di certezza dei rapporti giuridici, obbligando ad esempio i coniugi a trasmettere ai figli il primo cognome paterno e materno con la trasmissibilità solo del cognome paterno, sulla falsariga della normativa spagnola. Né possiamo tacere che neppure vediamo la *ratio* del testo in esame, allorché riflettiamo sulla circostanza che ben altre sono le disposizioni del codice civile che si pongono in contrasto con la Carta costituzionale, continuando a perpetrare una reale discriminazione tra uomini e donne e tra figli legittimi e naturali, segnatamente in materia ereditaria. Per questo motivo, ci sembra davvero risibile l'articolo 3 del testo in esame, che si illude (o ci illude) di cancellare ogni discriminazione soltanto perché sostituisce al termine naturale quello di figlio nato fuori del matrimonio. Si tratta di una denominazione ributtante e di una insensibilità umana inaccettabile, che perpetua più di prima un'intollerabile discriminazione a danno dei figli naturali. Si dirà: sei un figlio nato fuori dal matrimonio, quasi un figlio della colpa, e questo mi sembra un rimedio peggiore del male. La vera modifica da proporre, che qui si tace, è di richiedere che tutti i figli siano uguali anche dal punto di vista giuridico: che i figli sono figli, siano essi naturali, legittimi o legittimati. Occorre quindi abolire proprio le differenti denominazioni dei figli: i figli sono figli e basta, uguali da ogni punto di vista. In definitiva, si tratta di un provvedimento che richiede una profonda rivisitazione per ristabilire accanto al principio di eguaglianza quello della certezza dei rapporti giuridici, ma soprattutto è un provvedimento che va rivisto alla luce delle fondamentali ragioni dei figli, il cui stato giuridico ed è questa la questione fondamentale - non può subire discriminazioni di sorta.

termine: è stato iniziato l'esame del provvedimento sui DICO (è lì, se ne discute un po', un passo avanti, un passo indietro, avanti tutta, poi si va in piazza, poi si torna indietro); è stato incominciato anche il provvedimento sul testamento biologico, che in qualche modo attiene ad una delle certezze proprie del diritto, la disponibilità della vita e i confini della libertà.

- della discriminazione; questo è il nuovo tabù, il nuovo divieto di incesto, la nuova frontiera a cui tutti devono in qualche modo inchinarsi:

manifestazione di sudditanza culturale, ma anche un appiattimento di tutte le diversità e di tutte le convenzioni possibili, per cui vale solamente il principio dell'autodeterminazione, della libertà

principio costituzionale. Cosa c'entra questo con il provvedimento in questione? Certo, se il provvedimento viene motivato dalla necessità di eliminare qualunque forma discriminativa, in particolare,

secondariamente, quello dell'attribuzione del cognome paterno ai figli, su questa frontiera passa un progetto politico di scardinamento dell'identità, del diritto

stabilimento di regolazione dei rapporti familiari, soprattutto a livello maschile, e come secondo momento l'invidia del pene a livello della crescita femminile. Questo allora dovrebbe essere vietato:

Mettiamo Freud tra i libri proibiti, così come fece un regime ben preciso, che bruciò i libri di Freud per altre motivazioni,

uno sviluppo psicologico che è stato evidenziato, che fa proprio di questa differenza di genere un elemento non di disordine, bensì di ordine e di armonia, non si capisce perché si continui a negare il valore della storia, quindi della continuità e, anche, della trasmissione di determinati princìpi, a meno che non si voglia dire che,

il motivo della gentilezza, il motivo dell'armonia o anche del romanticismo, perché anche questa è una discriminazione di genere.

siamo stati abituati dalla medicina e dalla storia a considerare i generi sessuali come due, mentre abbiamo sentito, in Aula, parlare di discriminazione di genere, di identità di genere come determinata sulla base di un accesso o di una volontà individuale, per cui abbiamo appreso che ci sono addirittura sei generi diversi. Questo non appare nell'ecografia, in cui i generi sono necessariamente due; questo non discrimina poi sulla libertà di orientamento sessuale o di erotismo, come uno voglia sceglierlo.

È per questo che noi, non solo non possiamo condividere, ma rigettiamo il provvedimento in questione. In merito all'identità e all'attribuzione del cognome ai figli,

pensiamo che in queste radici del diritto di famiglia romanistica ci siano degli elementi che non debbano essere dimenticati. Non possiamo dimenticare che c'è stata una certezza di diritti affermata; non possiamo dimenticare che in qualche modo trasmettiamo un elemento di sicurezza, facendo passare il cognome

aveva una motivazione di eguaglianza; trasmettevamo un'eguaglianza e una certezza nei rapporti giuridici che con questo provvedimento andiamo fortemente a minare. Andiamo fortemente a minare il senso della storia e dell'appartenenza; noi crediamo che non si possa giocare con la certezza delle proprie radici e della propria identità. Oggi, la principale patologia sociale che cogliamo anche nell'ambiente medico è il difetto, la voglia

che manca all'interno della famiglia. Non c'è la necessità di creare personaggi da operetta; a me vengono in mente Zagor

che si vada a minare continuamente l'identità paterna e la certezza di ruoli che sono connessi

Il padre accetta i figli non in modo incondizionato, come fa la madre, ma se rispondono anche alla legge. Il principio della legge viene trasmesso dal padre e dall'unione del maschile e del femminile, che è dato appunto dall'unione tra un uomo e una donna e che fa parte di tutta la nostra storia psicologica, dei nostri archetipi (luna, sole e quant'altro), in 2000 anni di storia, si è generato l'equilibrio. Il polo dialettico dell'amore incondizionato della madre e dell'amore condizionato dell'uomo ha generato la tenerezza

ci affrontiamo, parlando di quanto manchi in questa società e della necessità di una cultura condivisa. Ma come possiamo

perché hanno applicato la norma del passaggio dei cognomi? Piuttosto, non riteniamo che compito della legge sia anche un'ordinata trasmissione di certezze e d'identità condivise? come possiamo condividere una storia, quando questa nasce in qualche modo da un elemento di rivendicazione?

consegnare al futuro, sempre e comunque, la storia passata. La tradizione è scegliere nel passato quanto deve essere consegnato alle generazioni future e, in qualche modo, deve essere mantenuto come un valore. La storia familiare e la certezza della propria identità di genere, la certezza della propria identità familiare: quanto può valere oggi la certezza di alcuni elementi condivisi, il cognome, le fotografie, gli oggetti? Ecco, noi vogliamo mettere in discussione forse tutto questo per un protagonismo forse esagerato, per il nuovo totem e tabù che è la discriminazione, ogni forma di discriminazione? Credo, colleghi, che il monito della Lega Nord sia quello di non togliere certezze, di valorizzare la differenza, di non considerare

il provvedimento che oggi stiamo discutendo è di grande delicatezza e importanza perché incide su due aspetti fondanti del convivere civile: da un lato, il sistema dei rapporti all'interno di quel nucleo sociale di base che è la famiglia, dall'altro, l'identità del nascituro. Di fronte al grande dibattito che avviene in questi mesi sul tema della famiglia, con questa scelta precisiamo non solo il nome, ma anche l'identità di questo nucleo sociale e, senza metterne in discussione l'unità e la funzione, si comincia a dire, laicamente, che questi caratteri si realizzano solo se sussistono parità e libertà. La denominazione familiare secondo il cognome del marito è un retaggio ormai superato dalla condizione che la donna ha acquisito nella società e nel lavoro ed è giusto, e forse tardivo, il riconoscimento di questo stato di cose. Affermare nel codice civile che ciascun coniuge mantiene, dopo il matrimonio, il proprio cognome, può sembrare piccola cosa, ormai consolidata dalla realtà, come dimostrerebbe il fatto, richiamato già nel dibattito e nella relazione, che negli atti ufficiali si utilizza il codice fiscale che notoriamente non muta con il matrimonio. Ma non si tratta affatto di piccola cosa: si tratta invece di riconoscere che la donna, nel matrimonio, sta con pari dignità e poteri rispetto al coniuge. È una piccola rivoluzione che oggi certifica il ruolo delle donne nella società. Tanta strada deve essere ancora fatta, però, per superare le discriminazioni che ancora appesantiscono la condizione delle donne nel nostro Paese. Basti pensare al fatto che la rappresentanza dei cittadini in questa stessa nostra Aula è ancora largamente maschile o alle altre discriminazioni, che le donne subiscono sul lavoro e nello sviluppo delle proprie carriere.

Ma oggi segniamo un importante risultato. Altrettanto rilevante di quella precedentemente indicata, è la scelta di dare logica conseguenza nell'assegnare i nomi ai figli. Sono state proposte diverse soluzioni per dare continuità al ruolo che la donna svolge nel dare la vita ai figli. Alcuni hanno proposto il doppio cognome obbligatorio, altri il solo nome della madre. Un dibattito come questo, anche per la sua delicatezza, deve essere affrontato senza atteggiamenti ideologici, senza asserzioni pregiudiziali, ma con il principio del dubbio e la capacità di ascolto. Io credo che sia necessario riconoscere il rapporto prioritario e privilegiato che la madre e il bambino hanno; tuttavia, la scelta di assegnare solo il cognome della madre non solo andrebbe contro l'idea della parità tra i generi, ma riconoscerebbe, forse erroneamente, solo quell'unico rapporto nel complesso sistema che si instaura dentro una famiglia. Così come l'idea che si obblighi all'assunzione di entrambi i nomi ha un sapore di anonima uniformità che non tiene conto delle differenze. Noi abbiamo in mente la famiglia come libera scelta di soggetti autonomi. È da qui che dobbiamo ripartire, dall'autonomia e dalla libertà. Per questo ci convince che il nome da dare ai propri figli, al frutto della propria libera scelta, sia una scelta libera tra i coniugi. È stato affermato da alcuni che questo provvedimento metterebbe in discussione l'unità della famiglia. Al di là della strumentalità del momento, non riusciamo a cogliere, nelle sue scelte di libertà, elementi che scardinino quel nucleo sociale, a meno che non si ritenga che ci sia una primazia maschile da riaffermare. L'ipotesi che una coppia decida di dare al proprio figlio il cognome della madre non mette in discussione l'idea della famiglia, bensì quella concezione distorta che si sviluppa solo intorno alla figura paterna. Oggi per fortuna non è più così. Le donne rivendicano il loro posto nella società a pieno titolo e rivendicano l'unicità femminile che si realizza nell'atto della nascita. In questi mesi autorevoli terapeuti hanno sollevato obiezioni prevedendo un futuro a fosche tinte. Hanno affermato che la scelta di chi deve dare il nome ai figli provocherà litigi e incomprensioni tra i genitori e che si creerà una perdita della linea genitoriale per arrivare a proporre di tenere come primo cognome quello paterno in tutti i casi. Si devono rispettare le opinioni degli scienziati e degli operatori, ma non vorremmo che la scienza fornisse alibi alla misoginia. Vorremmo, invece, affermare che ogni famiglia è un nucleo di soggetti liberi e autonomi che possono anche scegliere di avere figli e se ne assumono la responsabilità. Proprio in ragione di questa idea, la continuità della linea genitoriale paterna è uno degli elementi che configurano l'identità dei cittadini di domani, ma non certo quello più determinante. Un ultimo elemento di soddisfazione è la ridenominazione dei figli nati fuori del matrimonio. Si elimina così una discriminazione grave e si da completezza al percorso avviato fin dalla Costituzione. Il codice civile del 1942, emanato quindi prima della Costituzione del 1948, determinava con le sue norme una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali, sacrificandone diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani. La Costituzione, invece, non solo garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, ma impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela compatibile con quella della famiglia legittima. Resta allora a noi legislatori la responsabilità di consentire al Paese l'ultimo passo: attribuire, cioè, il diritto ai figli nati fuori del matrimonio di avere dei parenti, degli zii e dei nonni, dal punto di vista sia affettivo che legale ed economico. Con la speranza che tale questione possa essere affrontata rapidamente e l'augurio che il buon punto di equilibrio raggiunto in Commissione circa il disegno di legge in discussione possa essere confermato dall'Aula, siamo consapevoli che oggi si segna un risultato importante per affermare il ruolo delle donne nel nostro Paese e per dare attuazione a quel principio di pari dignità che la Costituzione prevede e sancisce.

avrei piacere innanzitutto che si rilevasse che su questa vicenda, di notevolissimo rilievo sociale, non vi è alcuna attenzione diffusa. Nel corso

Sta di fatto che una questione che riguarda 56 milioni di italiani, dunque tutti gli italiani (raramente il Parlamento discute provvedimenti che riguardano tutti gli italiani), è sostanzialmente ignota agli italiani. Questo è il primo punto da considerare. Non ritengo che siamo in ritardo, in ritardo, né che improvvisamente abbiamo deciso di occuparci di questa vicenda perché, come è stato scritto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, come si è detto in alcuni interventi e come è certamente il caso, questa materia è stata già oggetto di proposte di legge nella scorsa legislatura

e un insieme di interventi internazionali di altra natura ha posto all'attenzione la questione del rapporto marito-moglie, uomo-donna, genitori-figli. Tale la questione di fronte alla quale ci troviamo: ci troviamo: esiste nel nostro ordinamento costituzionale una definizione del rapporto genitori-figli che impone di avere una soluzione di un tipo anziché di un altro, oppure no? Il Parlamento, in altri termini, è in grado di poter fare qualunque legge ritenga di voler fare o è costretto, per Costituzione, a farne soltanto un tipo? Non pretendo che la mia opinione sia comune

non una somma di soggetti individuali. Questo il punto fondamentale che, a mio giudizio, rende impossibile una qualunque disciplina legislativa che tratti la questione del cognome dei figli come se si trattasse di una questione individuale. La questione è collettiva: è collettiva: riguarda la famiglia in quanto tale o certamente i genitori in quanto tali. Questa la ragione per la quale non possiamo fare riferimento ad altri Paesi stranieri, come se esistessero Paesi nei quali questi fatti avvengono al di là della decisione. Dobbiamo considerare che nel nostro ordinamento costituzionale, non per un fatto giuridico, ma per un fatto di straordinario rilievo politico-sociale, l'ordinamento familiare non può essere stabilito dal Parlamento secondo un criterio che prescinda da quelli che ritengo essere i vincoli della Costituzione. Si tratta di una questione che oggettivamente, in termini di studi sociologici e filosofici, è stata oggetto di discussione da almeno quarant'anni a questa parte, attraverso la questione del dibattito sul genere:

tra genitori e figli, ma un rapporto legato all'evolversi della cultura, dei rapporti sociali. È un fatto, cioè, che può essere cambiato con il mutare dei costumi sociali. Questo non ritengo sia conforme all'ordinamento costituzionale. Questo spazio di libertà del Parlamento nazionale non ritengo che esista, non per cattiveria, non perché lo dice la Conferenza episcopale italiana, non perché occorre essere, per così dire, clericali o religiosi ad altro titolo, ma perché nel nostro ordinamento costituzionale la questione fu una delle tre in ordine alle quali fu sancito il Patto costituzionale che regge il nostro Paese. Non è una questione di ordine, per per così dire, periferico; il Patto costituzionale, in virtù del quale il Parlamento non può legiferare su tutto ciò che vuole come gli aggrada - perché esiste un organo, chiamato Corte costituzionale, che ha il compito di dire che alcune leggi non si possono fare perchè la Costituzione lo vieta - fu sostanzialmente composto dalla riaffermazione dei princìpi di libertà individuali (cultura liberale classica), che ha dato vita a tutti i princìpi di libertà individuali (di associazione, di riunione, di corrispondenza, del dare vita a partiti politici e quant'altro); da una cultura di carattere collettivistico-sociale - parlo della cultura di matrice comunista, presente nella nostra Costituzione a vario titolo, soprattutto in materia economica - e da quella parte di cultura che si chiama cattolica, non in quanto clericale, ma laica, che afferma che è la persona, che precede lo Stato e non è un'affermazione che possiamo trovare in ogni Costituzione straniera - che concorre a dar vita a formazioni intermedie, una delle quali - una sola - viene individuata come radice costituzionale propria - la famiglia - con una sua specifica natura. È ovvio che questa specificità costituzionale non è lasciata, per così dire, in assoluta libertà, perché esiste in Costituzione il principio di eguaglianza. La Costituzione non scopre oggi il principio di eguaglianza. Essa prevede espressamente negli articoli 29 e seguenti che l'eguaglianza deve essere garantita all'interno della famiglia nei limiti dell'unità familiare. È la stessa Costituzione che non assume l'eguaglianza come valore generale, intorno al quale la famiglia può essere dissolta, ma il contrario: stabilisce che la famiglia deve essere ordinata secondo un criterio di eguaglianza tra i coniugi ed eguaglianza tra figli nati dentro o fuori del matrimonio. che la questione che abbiamo di fronte è sostanzialmente la prima: esiste o no nel Parlamento della Repubblica la convinzione che la famiglia è una formazione sociale?

il Parlamento può fare quel che ritiene, ma non può ignorare che la Costituzione afferma trattarsi di società naturale. Che significa società naturale in riferimento al rapporto genitori‑figli?

Anch'io colgo l'occasione per ringraziare il presidente e amico Salvi per aver concorso a condurre un dibattito su questo tema con estrema attenzione nel corso di molti mesi, ma noto, con sorpresa, che l'Aula è come se scoprisse il tema all'improvviso. Non si tratta di rinviare in Commissione il provvedimento, ma di capire di cosa stiamo discutendo. Il provvedimento approvato in Commissione giustizia è, a mio parere, contrario a questi princìpi costituzionali. A mio giudizio, questo provvedimento non parte dall'affermazione di un soggetto collettivo famiglia all'interno del quale esiste il rapporto genitori‑figli, ma afferma, ad esempio, che il rapporto dei genitori con i figli può portare ad attribuire

ignorare che si tratta di una legge che dovrebbe portare milioni di italiani, al momento del matrimonio, addirittura a decidere come si chiamerà il figlio, quale cognome dargli. Mi sembra voler innestare un elemento di conflittualità sociale particolarmente drammatico all'interno della vita, prevalentemente affettiva, di due persone che stanno per sposarsi. Ecco perché la questione deve essere risolta in termini automatici. Non può esservi incertezza su quale sia il cognome del figlio. In termini automatici si deve poter garantire o il mantenimento del modello patriarcale, che viene considerato superato contrario al principio di uguaglianza, oppure - a mio giudizio - si deve far sì che il principio di uguaglianza concorra a definire il modello familiare, ma non oltre. Il modello di uguaglianza non è il modello, per così dire, dell'indifferenza del cognome del figlio rispetto a quello dei genitori;

Ripeto, anche in questo caso può trattarsi di una questione sulla quale il nostro gradimento non è totale. Posso capire che ci possano essere idee diverse e in questo caso ovviamente si può tranquillamente dar vita a un ordinamento costituzionale diverso, ma fino a quando ciò non avviene mi sembra che il Parlamento sia vincolato in qualche misura

L'opinione di chi ritiene che sia necessariamente modificabile l'ordinamento del rapporto genitori-figli sulla base del mutare della cultura e della società una collega lo ha espressamente affermato e si tratta di un'affermazione giuridicamente significativa - e l'affermazione, della quale sono stato in parte protagonista, di chi ritiene che non vi sia una definizione di cultura che possa prescindere dalla definizione costituzionale dei rapporti fondamentali. L'Assemblea è chiamata a discutere di questo. Ho accolto con estremo interesse il riferimento fatto oggi dal presidente Salvi alla disponibilità ad una discussione anche più ampia che non in Commissione, lo dico con enorme piacere, perché questa materia, totalmente di origine parlamentare, non può che approdare ad un voto d'Aula costitutivo della natura del nostro Paese, che, per definizione, deve avere un larghissimo consenso parlamentare. Purtroppo, questo è mancato in Commissione; non è mancato per volontà ostruzionistica dell'opposizione: è mancato, secondo me, per una insufficiente valutazione complessiva delle cose; l'Aula è di fronte a questo problema, non al problema - che io non condividerei - di non discutere della materia, ma di fronte al problema di discutere della materia sapendo che di questo si tratta, non di un fatto banale e assolutamente periferico, ma di un fatto sostanziale dell'intera struttura del nostro Paese.

sospensive in modo da consentire l'avvio e la conclusione della discussione generale; al termine della discussione generale non vi è un accordo in base al quale il relatore deciderà che si torni in Commissione, ma prenderà atto del fatto che si vuole cercare un'intesa che vada al di là dello schieramento di maggioranza o di opposizione.

altrimenti, si vota sugli emendamenti e succeda quel che succeda. Non sono contrario all'ipotesi di rimanere in minoranza, ma è evidente che su una questione di fondo di questo tipo non si può far finta di non capire che siamo di fronte ad un elemento costitutivo della natura del nostro Paese

di libertà, a quel rapporto generale fra identità nazionale e identità di tipo diverso, perché questo fa parte della identità nazionale. Questo tipo di famiglia non è lo stesso che vi è nell'ordinamento svedese o in quello tedesco o in quello spagnolo o in quello austriaco:

il modello di tipo patriarcale, che si inserisca il principio di eguaglianza anche nella scelta del cognome dei figli e questo mi sembra opportuno e giusto. L'eguaglianza nella scelta del cognome dei figli significa che tra marito e moglie non deve esserci un'assoluta precedenza, ma non credo possa significare che vi sia l'indifferenza della genitorialità congiunta. Questo è un problema molto serio, sul quale, al termine della discussione generale, sarò molto lieto di conoscere l'opinione del Presidente della Commissione. Non c'è una richiesta, da parte del Capogruppo dell'UDC, di rimettere il disegno di legge alla non vi è l'idea di andare in Commissione senza che la questione sia più discussa, ma vi è l'idea che quello che viene dalla Commissione non può essere oggetto di un'intesa. Alcune proposte contenute negli emendamenti presentati in Aula sono considerate valide, altre no, non ho capito bene; se si vuole cercare un'intesa occorre capire su che cosa si vuole discutere;

su qualche quotidiano, soprattutto quelli economici, dello stato di crisi del nostro Paese, della mancanza di competitività,

chi saprà affrontarla andrà avanti, chi invece non saprà affrontarla tornerà indietro. L'Italia ha dei nodi strutturali pesantissimi,

neanche così fondamentale dal punto di vista ideologico, come la possibilità di cambiare il cognome degli individui.

essendo già sotto pressione, perché da più parti viene segnalato che il Parlamento, e in particolare il Senato, lavora poco (e qui ci sono i numeri

più impegnativo sul piano mediatico, che vuole regolamentare le coppie di fatto. È evidente che i due provvedimenti sono figli della medesima ideologia; è evidente che intendono attaccare e cambiare in radice il nucleo fondamentale della nostra società, la famiglia, così come finora concepita, cioè l'unione di un uomo e di una donna atta a procreare una discendenza.

il suffisso «son» svedese. Quindi, la necessità d'individuare la discendenza e dichiarare la propria appartenenza affonda nelle radici della nostra storia.

non c'è più proletariato, perché ormai è scomparso (almeno dalle nostre plaghe): egli definisce queste nuove masse che hanno a che fare con l'impero e la globalizzazione «la moltitudine».

paragoni pop - quella del film «Blade Runner»: un mondo in cui esiste una moltitudine senza punti di riferimento. È chiaro che, se questa è la concezione di chi oggi si sente ancora figlio del materialismo storico,

Qui nascono le contraddizioni, perché - come dicevo prima - la vostra maggioranza non è assolutamente coesa su tali temi. Si è stati costretti a cercare dei difficilissimi punti di incontro che, in realtà, non sono ancora stati trovati. Anche sotto questo punto di vista credo che la presentazione in Aula del disegno di legge sia assolutamente prematura. Perché? Ripercorriamo

Tutta la partita si è giocata in uno scontro maggioranza-opposizione all'interno della maggioranza stessa con, ad esempio, il ministro Bindi in grave difficoltà perché ha visto alcune proposte essere brutalmente bocciate dalla sua maggioranza. Alla fine si esce con questo testo che contiene

una possibilità di poter uscire da questa problematica, perché - ripetiamo - è una questione di natura ideologica. Pensiamo che questo sia un provvedimento, come dicevo poc'anzi, che fa parte del più vasto piano di attacco alla famiglia, non quella tradizionale

articoli 29, 30, 31 e 32 (cito a memoria e spero di non sbagliare) e ci sono delle chicche che derivano sempre dalla necessità di trovare faticosamente una sorta di compromesso fra le diverse anime della maggioranza. Cito la più clamorosa, contenuta all'articolo 2, per cui se i genitori sono d'accordo, bene, si sceglie il cognome fra l'uno e l'altro, ma se non sono d'accordo cosa si fa? Si tira a sorte! Pensate: il cognome, che è elemento costitutivo di un individuo, viene determinato attraverso l'alea. Mi domando se questa sia una soluzione seria. lo credo, ma non voglio ironizzare più di tanto. Ciascuno di noi tiene alla propria discendenza e al proprio patronimico: ebbene, domani questo individuo, in attesa di suo figlio, che magari nascerà in provetta, comunque vedrebbe il suo cognome discendere dal cielo tirato a sorte. Qui c'è il relatore, che probabilmente starà pensando ad altro, ma sarebbe interessante capire come possa nascere... di questo mi compiaccio e mi complimento con lei, senatore Salvi, ma dovrebbe poi dirci perché si è arrivati a questo...

dicevo, sarà interessante capire. Francamente, come individuo sarei molto seccato se il mio cognome dovesse essere determinato dalla dalla sorte. Sono contento di essere figlio di chi mi ha generato, di mio padre: quindi, sono molto contento di portare un nome che risale magari un po' in là nel tempo. La seconda questione

addirittura di morte - quindi, anche nel caso in cui magari c'era l'accordo, ma non è più possibile trovare i genitori - si tira a sorte. Francamente, mi pare una soluzione non molto dignitosa per un provvedimento di legge.

di un bambino o di una bambina? All'ufficiale dell'anagrafe, che lo farà magari in nome di una cultura sua propria, completamente lontana da quella del luogo in cui invece è nato

In ogni caso,